Comunico che in data 28 giugno 2023 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze:* «Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi» (781).

*(Az-IV-RE)*. Signor Ministro, la ragione per la quale sono qui ad interrogarla oggi è relativa alla situazione dell'ex hotel Astor di via Maragliano a Firenze. di un immobile che dal settembre 2022 risulta occupato da una settantina di persone. Da quel momento la comunità cittadina e tutte le persone che abitano nei dintorni dell'ex hotel hanno

in questo edificio si sono avuti una serie di incidenti anche molto seri. Nel mese di marzo i cittadini hanno denunciato una sorta di maxirissa con violenze con bastoni, bottiglie, scacciacani e quant'altro. Ancora peggio,

se una caduta dal terzo piano non è mai una bella cosa. In questa situazione già esplosiva si è verificato un

Della bambina non ci sono tracce e ci si chiede se questo episodio non si sia verificato anche a cagione del fatto che l'ambiente nel quale la bambina viveva non era certamente un ambiente sano. sano. Quando c'è un'occupazione, ai sensi dell'articolo 633 del codice penale, si possono verificare due fatti: o la Polizia giudiziaria, *ex* articolo 55 del codice di procedura penale, procede allo sgombero, oppure ci vuole un sequestro preventivo della procura della Repubblica;

l'ex hotel. Da notizie risulta che la Digos avesse più volte chiesto alla procura di emettere questo sequestro preventivo, perché erano evidenti i problemi di ordine pubblico, ma questa decisione della procura non era arrivata. Vorrei pertanto sapere da lei che cosa mi può riferire relativamente al ritardo nella decisione di sgomberare l'immobile e se il Ministero non ritenga che il caso della bambina scomparsa non dipenda anche dal fatto che tale decisione non è stata presa tempestivamente.

esclusivamente descrittiva e interlocutoria, perché quando vi è un'indagine in corso il Ministro della giustizia non ha poteri e non deve interferire con il procedimento giudiziario. posso soltanto descrivere quanto ci risulta dalle note che abbiamo acquisito. risale al 18 settembre 2022 l'occupazione di questo immobile per il quale la procura della Repubblica di Firenze, in data 30 settembre, ha iscritto un procedimento penale. Gli autori della condotta venivano compiutamente identificati nell'immediatezza dei fatti: si trattava in prevalenza di nuclei familiari composti anche da 11 soggetti minori degli anni diciotto, in gran parte di età infantile. Secondo quanto indicato dalla Polizia giudiziaria, l'immobile, che era già sede dell'hotel Astor, risultava da tempo in disuso e in stato di abbandono ed era stato oggetto di precedenti occupazioni. Con riferimento a tale immobile, si rilevava l'esistenza di plurimi procedimenti penali in relazione al reato previsto e punito dall'articolo 633 del codice penale, che l'interrogante ha citato, per fatti commessi tra il 2014 e il 2022. Il 17 novembre del 2022, d'intesa tra la procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze e il dirigente della Digos di Firenze, la situazione veniva continuamente monitorata e sottoposta a complessiva ricognizione per censire gli occupanti e i relativi nuclei familiari. In quella data erano in totale 54,19 dei quali minori degli anni diciotto, suddivisi in 17 nuclei familiari. In quell'occasione alcuni degli occupanti si impegnavano a lasciare l'immobile, le donne in gravidanza o con bambini manifestavano la loro disponibilità a trasferirsi in altri luoghi da individuare e la presa di contatto dei servizi sociali con gli occupanti e l'instaurazione di una relazione continuativa con l'offerta di supporto costituivano l'avvio di un percorso che appariva proficuo e utile per una ragionevole ricollocazione di questi nuclei. Senonché, in data 28 gennaio 2023 la procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze spediva l'avviso di conclusione delle indagini preliminari per il procedimento penale che ho citato prima e veniva emesso il decreto di citazione diretta con una prima udienza fissata per il 22 maggio 2024. Nel maggio del 2024, quindi, si celebrerà questo processo. Intervenivano poi dei fatti nuovi. In seguito a un tentativo di omicidio del 28 maggio 2023 all'interno di questo immobile, la procura di Firenze chiedeva informalmente alla Polizia giudiziaria di verificare se vi fosse interesse da parte della parte offesa a presentare una nuova querela. Il 10 giugno 2023, nell'immobile occupato, veniva rapita la minore, di cui non cito il nome, fatto per il quale veniva iscritto un procedimento penale in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione. Dopo la presentazione, il 14 giugno 2023, della querela ad opera del proprietario, veniva avviato un nuovo procedimento penale sempre ai sensi dell'articolo 633 nell'ambito di questo procedimento il 16 giugno 2023 veniva richiesta al giudice per le indagini preliminari l'adozione di un decreto di sequestro preventivo dell'immobile, provvedimento di coercizione reale che veniva emesso in pari data ed eseguito il 17 giugno 2023. Allo stato, secondo quanto rappresentato dalla locale procura, non sussistono elementi idonei a ritenere che il rapimento della minore possa essere in qualche modo ricondotto alla sua permanenza all'interno dell'immobile occupato.

voleva in realtà accendere una luce sull'indagine in corso, perché è giusto che prosegua così e anzi auspichiamo che la bambina sia trovata sana e salva. Il problema era sostanzialmente un altro, cioè comprendere per quale motivo il provvedimento di sgombero sia stato adottato dopo che una situazione che era evidentemente insostenibile è esplosa con questo caso, che naturalmente ha acceso l'interesse dell'opinione pubblica, perché la sparizione di una minore è un evento di una minore è un evento di una gravità massima e inaudita. Chiaramente la situazione, che era sconosciuta al grande pubblico, all'opinione pubblica nazionale, ma ben conosciuta da chi abitava nei dintorni dell'ex hotel Astor, Astor, è esplosa ed evidentemente è sembrato un provvedimento reattivo rispetto a un problema. La domanda è perché questo provvedimento, che è sembrato fondamentale il 17 giugno, non fosse stato assunto in precedenza. È successo qualcosa, ma la domanda è questo qualcosa si sarebbe potuto evitare se la decisione fosse stata presa prima. Questo è il punto, perché il problema - noi ne parliamo spesso e ci è capitato di interloquire anche in Commissione giustizia ovviamente l'obbligatorietà dell'azione penale mette i giudici davanti a un tale numero di stimoli e di possibilità di esercitare l'azione penale, che poi vanno fatte delle scelte. In questo caso si è scelto di non agire, perché forse si è ritenuto che ci fossero altre emergenze. Può anche esserci la responsabilità di una scelta, però, signor Ministro, la responsabilità della decisione si deve accompagnare anche alla responsabilità degli eventuali errori nella scelta. Questo è il vero punto della questione. La domanda era questa, ovviamente lei non mi ha potuto rispondere, quindi non posso dirmi soddisfatto della sua risposta, ma le sottopongo ancora una volta un problema di cui abbiamo già parlato.

Presidente, signor Ministro, ci risulta anche da notizie di stampa che sia stato firmato un importante accordo interistituzionale dal Ministero della giustizia e dal

Per un verso, sicuramente la recidiva non risolve; secondariamente, ma non da meno, dobbiamo attestare e prendere atto dell'inefficacia dei rimedi che sono stati adottati con i cosiddetti provvedimenti svuotacarceri (perdonatemi l'espressione). invece, ci troviamo di fronte a una nuova soluzione che è molto importante, perché se la rieducazione della pena avviene attraverso la possibilità di agevolare l'inserimento lavorativo e quindi l'inserimento sociale del condannato, andiamo incontro e rispettiamo la Costituzione e le stesse persone che subiscono una detenzione in carcere. A volte, infatti, il carcere da solo, senza altri strumenti, non educa. Signor Ministro,

Ci stiamo anche occupando, non soltanto del lavoro all'interno delle carceri, quanto della possibilità di trovare il lavoro dopo la scarcerazione del detenuto e in questo senso ci siamo già attivati attraverso varie fondazioni. Qui si inserisce questo accordo con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che ha lo scopo di promuovere, attraverso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, proprio l'inserimento lavorativo delle persone in esecuzione della pena detentiva. I dati sono abbastanza indicativi: le persone che vengono inserite in un percorso lavorativo all'interno del carcere e poi trovano un lavoro, una volta dismesse dall'istituto penitenziario, tendono alla cosiddetta recidiva zero, mentre le persone che in carcere non riescono a realizzare le proprie aspirazioni anche in senso lavorativo, una volta uscite, tendono a essere recidive. In quest'ottica, il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro hanno avviato una collaborazione per diffondere, favorire e semplificare le modalità di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi offerte ai detenuti. Collaboreranno, altresì, nel contribuire all'evoluzione del quadro normativo e giuridico nel rispetto dell'esigenza di favorire questo processo di reinserimento e valuteranno l'incremento dei percorsi di formazione, anche universitaria, e di riqualificazione professionale. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'accordo che è stato già firmato è stata prevista la costituzione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di un'apposita cabina di regia che sarà sotto la guida del sottosegretario di Stato alla giustizia con delega al trattamento dei detenuti, senatore Ostellari, con il compito di trasmettere periodicamente al Ministro della giustizia e al Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro risultati dell'attività svolta per la preparazione e l'adozione delle conseguenti iniziative. Questa per noi è una priorità. Lo ripeto per l'ennesima volta. Noi siamo garantisti, ma il garantismo va inteso in due modi: come enfatizzazione della presunzione di innocenza prima del processo e come certezza dell'esecuzione della pena dopo la condanna definitiva. L'esecuzione certa della pena, però, deve sempre tenere presente l'articolo della Costituzione che mira alla rieducazione e al reinserimento

Esprimiamo poi piena soddisfazione perché per lavorare su certi temi, soprattutto su alcuni molto articolati, occorrono co-progettazioni e cooperazione anche fra gli stessi enti, fra il pubblico e il privato e ciò vale anche per la giustizia e lei, signor Ministro, ci ha dimostrato infatti che

Ministro, il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Milano ha presentato un *report* sulla situazione in cui versa l'istituto penale per i minorenni «Beccaria» di Milano, nel quale si evidenzia l'aggravarsi delle già precari condizioni dell'istituto da dove, com'è noto, lo scorso Natale sono evasi sette detenuti. Si legge nel *report* che la situazione giovanile è estremamente preoccupante e i ragazzi che arrivano hanno delle modalità relazionali molto aggressive, spesso con problematiche dovute, non solo alla condotta, ma anche legate all'uso di droga e problemi psichiatrici. Trovare posto in luoghi alternativi non è facile. A oggi ci sono sette provvedimenti di collocamento in comunità, ma non si trovano posti perché le comunità rifiutano di accoglierli Infatti, ad oggi, sono ben settanta i dinieghi registrati. Fra i motivi addotti per tali dinieghi ci sono la carenza di spazi, le forti problematiche presentate dai ragazzi e in particolare l'essere molti di loro minori non accompagnati, oltre alle difficoltà nel trovare gli educatori, che notoriamente sono pagati con stipendi assolutamente inadeguati rispetto al delicatissimo ruolo che sono chiamati a svolgere. Nel *report* del Garante, inoltre, si evidenzia la particolare criticità delle condizioni di vita dei ragazzi in isolamento che, come si può leggere, pranzano coi piatti sulle ginocchia per l'assenza di tavolini nelle celle, dove anche l'utilizzo di tavole di plastica o a ribalta non risulta adeguato per ragioni di sicurezza. di sicurezza. Relativamente al personale, il *report* del Garante evidenzia come ogni anno la maggior parte del personale, che spesso è giovanissimo, chieda il trasferimento nel luogo di origine o un luogo più vicino, con richieste che comportano un continuo *turnover* del personale; alle emergenze che si vengono a creare si risponde di volta in volta facendo ricorso a rinforzi estemporanei per brevi periodi; è la mancanza di un progetto educativo, oltre alla mancanza ormai decennale della stabilità nella figura del direttore e del comandante degli agenti di Polizia penitenziaria, che reca un grave nocumento al funzionamento dell'istituto; vi è anche la questione degli spazi. Per carità, abbiamo visto che finalmente viene inaugurato un nuovo padiglione dopo tanti anni. Questa è una buona notizia, ma gli altri problemi restano. Chiediamo quindi di sapere quali iniziative necessarie e urgenti il Ministro intende intraprendere per stabilizzare anzitutto la direzione

ed è inutile che spieghi quanto queste siano limitate. Comunque, le notizie che vi do sono asettiche e rispecchiano, io credo, l'impegno di questo Governo per colmare le suddette lacune. È stato stipulato un accordo - il 26 gennaio 2023 - tra l'azienda sociosanitaria territoriale Santi Paolo e Carlo della Regione Lombardia e il Ministero della giustizia che ha ad oggetto la graduatoria del concorso pubblico a tempo pieno e indeterminato di collaborazione di personale sanitario ed educatore professionale di categoria D. Nello specifico, sono stati assunti quattro funzionari di professionalità pedagogica, tre dei quali hanno preso servizio in data 12 aprile 2023. Il prossimo prenderà servizio il 20 luglio. È in corso di svolgimento il concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo di 773 unità, di cui 360 funzionari di professionalità pedagogica. Per quanto riguarda il Corpo di polizia penitenziaria si fa presente che l'organico dell'istituto penale Beccaria è stato determinato in 71 unità

Per quanto riguarda i collocamenti in comunità, bisogna specificare che, come lei stesso ha rilevato, di fronte all'elevato numero di richieste da parte dell'autorità giudiziaria, le strutture comunitarie disponibili sul territorio non riescono a garantire una sufficiente ricettività. Si rappresenta - lo voglio dire da ultimo - che in data 14 settembre 2022, in sede di Conferenza unificata, è stato sancito l'accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali che è rivolto alla costituzione di comunità sperimentali di tipo sociosanitario, a elevata integrazione sanitaria, per l'inserimento di minori e giovani adulti con disagio psichico e problematiche di dipendenza. Il percorso è lungo e difficile, però vi voglio assicurare che fa parte proprio delle nostre priorità, perché se la criticità negli istituti penitenziari è già elevata quella che riguarda gli istituti minorili deve avere una priorità alla quale prestare un'attenzione ancora maggiore.

Le dico anche che non attribuiamo a lei le responsabilità annose della situazione del Beccaria e delle carceri minorili. Però, nei giorni scorsi, il 12 giugno, è stato il cappellano del carcere, don Claudio Burgio, a dire testualmente che la situazione è persino peggiorata dai giorni dell'evasione. I lavori sarebbero terminati, ma i locali verranno assegnati ad ottobre, così come il nuovo direttore. I rinforzi di Polizia penitenziaria non sono arrivati e gli educatori in più erano, a quella data, soltanto due. Rimane drammaticamente carente - lo ha ammesso anche lei - la comunicazione tra carceri minorili e rete di accoglienza. Il problema non riguarda solo il Beccaria; a Nisida la situazione è altrettanto drammatica, toccata con mano nei giorni scorsi da una delegazione, anche del nostro partito. Ministro, una responsabilità gliela attribuiamo: lei non ha dato segnali di direzione del trattamento dei minori che si trovano nelle carceri e dovrebbero trovarsi lì per un reinserimento. Invece di introdurre temi divisivi, che tra l'altro rischiano di minare la lotta alla corruzione, applichi le riforme che le abbiamo lasciato in eredità: la riforma Cartabia prevede importanti iniziative per la messa alla prova e la giustizia riparativa per i minori. Si attivi - lo diciamo davvero - per accelerare l'assunzione di magistrati, anche nei tribunali dei minori, per stabilizzare i 16.000 addetti degli uffici del processo, per cercare di aumentare il personale, applicare le riforme e non divagare con temi divisivi. Infine, sostenga il lavoro delle comunità di accoglienza per favorire il reinserimento e il lavoro di questi poveri giovani, spesso emarginati, che stanno lì anche impropriamente. Sulle carceri ho davvero finito. Perché non ha ascoltato i nostri ripetuti appelli per non far tornare a dormire in carcere i detenuti semiliberi che da due anni lavoravano e dormivano fuori? Invece sono rientrati; altro che lotta al sovraffollamento. Perché non garantire la telefonata quotidiana dei detenuti alle loro famiglie? Sarebbe un fatto importante. Ecco perché non siamo soddisfatti, Ministro. Lei si proclama - e certamente lo è nel suo intimo - garantista, però mi creda: cerchi di iniziare dai poveri cristi e non dai colletti bianchi ad essere garantista.

Signora Presidente, illustre signor Ministro, da alcuni anni in tutta Europa, ma anche in Italia fortunatamente, gli investimenti sulla sfera del digitale per l'implementazione dei servizi sono cresciuti in via esponenziale, anche nelle strutture pubbliche e nelle articolazioni centrali e periferiche dello Stato, con specifico riferimento al complesso comparto dell'amministrazione della giustizia. Le restrizioni dovute alla drammatica emergenza pandemica, con la moltiplicazione dei servizi telematici e dei cosiddetti sportelli virtuali che erano finalizzati a ridurre al minimo gli accessi fisici presso strutture, università, tribunali Ministeri e uffici, da limite si sono trasformati in una straordinaria opportunità per la Nazione e hanno prodotto, quindi, un'accelerazione inarrestabile verso il futuro. In questo senso, anche i servizi di cooperazione informatica appaiono sempre più fruttuosi, purché naturalmente vengano realizzati in una cornice di sicurezza, in un trasferimento massivo di informazioni e di dati particolarmente sensibili. Per questo gli osservatori più attenti, in modo particolare gli operatori in ambito giuridico, hanno accolto con grande interesse ed attenzione, nei giorni scorsi, l'intervenuta sottoscrizione di una

del precetto normativo di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, che consenta di accedere direttamente, da parte degli ufficiali giudiziari, alle banche dati dell'amministrazione finanziaria. Siamo quindi a interrogarla, ai sensi del Regolamento, per avere informazioni di maggior dettaglio, *in primis* sull'orizzonte temporale lungo il quale questa convenzione dovrà dispiegare i suoi effetti in secondo luogo, sulle garanzie predisposte dal suo Ministero sulla sicurezza del trattamento dei dati trattati. Soprattutto, interessa comprendere quali riflessi pratici si proponga il Governo e quali vantaggi e benefici si prevede che la convenzione possa determinare per gli operatori del diritto, da un lato, e soprattutto per i cittadini tutti. la risposta è più facile e finalmente possiamo dare buone notizie. Quando parliamo di carceri, si parla sempre di un fardello di dolore, ma in questo caso, per fortuna, possiamo parlare di qualcosa di positivo e di utile anche per la nostra economia. Sono dati tecnici, quindi li riferirò così come li ho ottenuti, dopo un *excursus* estremamente accurato. Questa convenzione, stipulata il 23 giugno tra il Ministero della giustizia e il direttore dell'Agenzia delle entrate, con l'approvazione del Garante per la protezione dei dati personali, consente agli ufficiali giudiziari di accedere alle banche dati dell'amministrazione finanziaria, così da rendere agevole la ricerca telematica dei beni da pignorare. È una cosa quasi rivoluzionaria. Si tratta di beni da pignorare, ovviamente, in seguito alla richiesta del creditore, ovvero da sottoporre a procedura concorsuale, in questo caso su richiesta del curatore. Prima della stipula di questa convenzione, in forza dell'articolo 155-*quinquies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che era stato inserito nella legge del 2014, era previsto che, in mancanza delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto, il creditore istante potesse ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni in esse contenute. Con questa Con questa novella dell'articolo 155, introdotta nell'ottobre 2022, è stato previsto che, a decorrere dal 28 febbraio 2023, fosse l'ufficiale giudiziario ad attestare che l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile per il mancato funzionamento delle strutture tecnologiche. Ecco perché, a seguito della stipula della convenzione del 23 giugno 2023, gli ufficiali giudiziari possono utilizzare direttamente il servizio di accesso alle banche dati dell'amministrazione finanziaria nell'ambito dei propri compiti di ufficio, al fine di acquisire tutte le informazioni utili a individuare i beni da sottoporre a esecuzione forzata nell'ambito delle procedure sia immobiliari sia mobiliari, nonché nell'ambito di quelle concorsuali. In dettaglio, l'ufficiale giudiziario può richiedere all'Agenzia delle entrate l'accesso alle sue banche dati in relazione a soggetti, che siano il debitore esecutato o sottoposto a procedura concorsuale, per i quali è stata presentata istanza da parte di un creditore in possesso di un titolo esecutivo e del precetto, in seguito alla specifica autorizzazione del presidente del tribunale. A quel punto, l'Agenzia delle entrate, verificata la regolarità della richiesta, invierà la risposta con le notizie al sistema informatico del Ministero della giustizia. Questo permetterà una più rapida verifica sui beni di proprietà del debitore, consentendo al creditore di velocizzare il recupero del credito vantato. Il vantaggio consisterà nella certezza e nella celerità della ricerca di beni da pignorare, assicurando quindi un *iter* più spedito nelle esecuzioni dei provvedimenti del giudice in materia civile. Ovviamente, gli accessi alle banche dati dell'amministrazione finanziaria e le relative richieste resteranno tracciati. Questo secondo me è un passo molto importante ai fini dell'accelerazione della certezza dei rapporti economici che derivano da quelli giuridici, in riferimento ai quali - lo ripetiamo ancora una volta - la lentezza della nostra giustizia è giudicata così critica dagli investitori stranieri che l'investimento in Italia risulta per loro in questo momento

in primo luogo - me lo consentirà - sotto il profilo delle garanzie, quelle di necessaria riservatezza, previste dalla convenzione e peraltro validate dal Garante per la protezione dei dati personali, in merito al tracciamento e alla registrazione degli accessi e delle operazioni, che consentiranno sicuramente le successive verifiche di correttezza e di legittimità, come anche con riferimento alle procedure di gestione delle eventuali anomalie che dovessero risultare. Siamo poi soddisfatti anche delle sue precisazioni in punto di strumenti individuati dalla convenzione, sempre più orientati alla semplificazione delle procedure e alla celerità degli accertamenti: un accesso sempre più snello per la ricerca di beni e crediti da sottoporre ad esecuzione un accesso alle banche dati più diversificate (anagrafe tributaria, archivio dei rapporti finanziari, informazioni degli enti previdenziali). Questo sia su richiesta di chi vanti un credito e sia naturalmente in possesso di un precetto o di un titolo esecutivo, sia su istanza del curatore che debba individuare i beni da sottoporre a procedura concorsuale. Siamo convinti dei possibili benefici da lei preventivati, ma quel che più conta, signor Ministro, è che noi siamo soddisfatti delle sue risposte per la filosofia che ispira questa convenzione, quella della sempre maggiore certezza delle posizioni giuridiche, che rimane uno dei pilastri fondamentali e irrinunciabili di uno Stato di diritto. Grazie ancora, signor Ministro, e buon lavoro.

contemporaneo offre tante possibilità e tante opportunità, ma dietro l'angolo ci sono tante insidie lungo il percorso della crescita dei nostri ragazzi. Accade quindi molto spesso - lo sentiamo e lo leggiamo dalla cronaca - che queste sfide diventino sfide diventino un peso enorme per i nostri ragazzi, con un sovraccarico di ansia che non si riesce a superare. Non ne hanno assolutamente colpa i nostri ragazzi; l'unica colpa può essere quella anagrafica, di essere giovani e di non avere una struttura tale da riuscire a far sopportare loro questo percorso di

cardine del mandato del Governo, in particolare del ministro Bernini, e cioè il benessere psicologico delle studentesse, degli studenti e dell'intera comunità universitaria. Le varie inaugurazioni degli anni accademici a cui ha partecipato, spesso anche in prima persona, il ministro Bernini sono state un'occasione di confronto con centinaia di studenti e in molti, purtroppo, hanno rilevato - come diceva anche l'interrogante - di aver sofferto un disagio psicologico, ansia da prestazione e paura di non farcela. Il benessere dei nostri studenti richiede un impegno assoluto e corale; è un'esigenza che dobbiamo garantire insieme alle istituzioni, alle università e naturalmente alle famiglie. Come correttamente ricordato dal collega Damiani, con la recente conversione del decreto-legge pubblica amministrazione è stato introdotto nelle AFAM e nelle università il docente delegato, che è dedicato al coordinamento e al monitoraggio di tutte le iniziative legate al supporto e al benessere psicologico degli studenti. È un ulteriore passo in avanti per rispondere a un'esigenza concreta di sostegno, con nuove modalità di ascolto e di supporto per il benessere della comunità universitaria. Il Ministro dell'università e della ricerca si è attivato per fare di più, in modo da dare risposte strutturate e durevoli nel tempo. Per questo motivo, è stato previsto - nel riparto del fondo di finanziamento del 2023 - uno stanziamento di 35 milioni di euro a sostegno dei programmi di ateneo per il potenziamento dei servizi a favore degli studenti, tra cui quelli finalizzati a promuovere l'inclusione, nonché all'attivazione e al potenziamento di servizi di supporto e sostegno psicologico specifici. Ad essi è intenzione del ministro Bernini aggiungere ulteriori 5 milioni di euro per le medesime finalità, per un totale di 40 milioni. Altri 13 milioni di euro del fondo sono destinati poi a interventi di sostegno dedicati agli studenti con disabilità, con un incremento di 5 milioni rispetto allo scorso anno. L'università non si può ridurre al sostenimento degli esami o a una corsa alla pur importante corona d'alloro. L'università è anche un reticolato di rapporti umani, fondamentale per conseguire un bagaglio di esperienze e di strumenti utili per la vita. È questo che auguriamo e che si cercherà in ogni modo di assicurare.

per il suo tramite mi rivolgo al Ministro dell'università e della ricerca. Stiamo vivendo un momento drammatico di carenza di personale sanitario, in particolare di personale medico specialista. Questo succede anche perché l'Italia non ha mai avuto una struttura di programmazione del fabbisogno di specialisti in ambito sanitario. E allora nella legge di bilancio del 2020 abbiamo approvato una norma che istituiva proprio una tecnostruttura - tra osservatorio, scuole di specializzazione e Agenas - che serviva a programmare il fabbisogno di specialisti.

se avesse in programma di far partire la struttura e la Ministra mi rassicurò sul fatto che a breve la struttura sarebbe diventata operativa. Un mese dopo, però, è stato ritirato l'interpello che prevedeva l'incarico del direttore generale di quella struttura. Inoltre, l'articolo 9 del decreto-legge n. 44 del 2023

a ciò, ci sono state altre due norme in ambito di formazione specialistica: il decreto-legge n. 51 del 2023, il cosiddetto decreto *omnibus*, che ha anticipato al secondo anno l'assunzione dei medici in formazione specialistica, e il decreto interministeriale n. 138 del 2023, che ha previsto una sensibile riduzione dei volumi dell'assistenza minimi per l'accreditamento delle scuole di specializzazione.

delle scuole di specializzazione, se non si intenda invece ripristinare quella struttura che era voluta dal Parlamento e che aveva in dotazione 3 milioni di euro all'anno, o se si intenda invece trasformare una di queste due nuove direzioni in una struttura dedicata esclusivamente alla formazione, e se non si ritenga che questo abbassamento degli *standard* formativi previsti per l'accreditamento delle scuole di specializzazione, così come la possibilità di assumere i medici in formazione già dal secondo anno, sia invece un rischio per la qualità della formazione dei nostri medici in formazione specialistica.

per l'interrogazione. La diffusione della pandemia da Covid-19 ha reso quanto mai evidente la necessità di personale medico qualificato e numericamente adeguato alle esigenze della nostra popolazione. Per questo, la valorizzazione e il sostegno del percorso di formazione delle professioni mediche con azioni mirate, volte a consentire di garantire *standard* qualitativi elevati e competitivi a livello internazionale, costituiscono obiettivi prioritari per il Governo e naturalmente anche per il ministro Bernini. L'obiettivo è quello di adottare una politica organica per la programmazione sanitaria composta da interventi sull'accesso ai corsi in medicina e alle scuole di specializzazione medica. Sull'acceso programmato ai corsi in medicina è stato avviato presso il Ministero un gruppo di lavoro già dal gennaio scorso, che ha coinvolto il Ministero della salute, esperti del mondo accademico, la Conferenza Stato-Regioni ed esponenti degli ordini professionali interessati, per definire il fabbisogno dei medici e adeguare le capacità e l'offerta potenziale del sistema universitario. Il lavoro svolto è stato attento e ambizioso e ha consentito di adeguare le capacità e l'offerta potenziale del sistema universitario in via transitoria rivedendo i meccanismi di programmazione degli accessi e di porre solide basi per un ampliamento a regime. Nel solco di questo lavoro proficuo, è intenzione del Ministero promuovere un'iniziativa analoga anche per l'accesso alle scuole di specializzazione di area medico-sanitaria, considerata la stretta consequenzialità con l'aumento del numero dei posti disponibili alla facoltà di medicina. Alla formazione specialistica universitaria nel settore sanitario saranno dedicati gli sforzi del Ministero anche monitorando la qualità della formazione degli specializzandi, affinché la professione medica sia svolta con competenza e professionalità. In questo senso, l'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica sta completando il processo di accreditamento delle scuole e ciò avverrà in tempo utile affinché i candidati del concorso indetto lo scorso maggio possano effettuare le scelte delle sedi e delle scuole attivabili dal prossimo autunno. La revisione delle strutture ministeriali oggetto dell'interrogazione è funzionale a garantire una migliore gestione di tutte le competenze attribuite al Ministero. Agli alti studi medici sono rivolti ancora ulteriori sforzi e tranquillizzo l'interrogante, della qualità del sistema universitario e sanitario sarà al centro dell'agenda politica del ministro Bernini. In conclusione, la ristrutturazione complessiva del Ministero ancora di più assicurerà coerenza ed efficienza a un'area altamente strategica per il nostro Paese.

una struttura che serviva proprio a programmare il fabbisogno specialistico. Perché cancellarla riportando le competenze a una direzione del Ministero? Il Ministero già oggi aveva l'obbligo di monitorare l'Osservatorio scuole di specializzazione, ma senza una struttura dedicata che si coordini con Agenas, questo non è successo. Abbiamo visto - e inchieste

e mettere al centro la qualità della formazione, è necessario investire e qui gli investimenti ci sono, perché tre milioni di euro all'anno erano dedicati proprio a questo, alle *site visit*, agli accreditamenti,

specializzazione dalla rete formativa significa rischiare che facciano una formazione che non è più di qualità, perché oggi quei volumi formativi che prima erano garantiti da una rete verranno erogati da una sola struttura e quindi si ridurrà la varietà, che invece è fondamentale per una formazione specialistica di qualità.

Grazie,

La prima domanda che ci facciamo è che fine abbiano fatto tutte le promesse che ha fatto il ministro Musumeci, quei tavoli settimanali con la Regione e con i sindaci del territorio Abbiamo accettato le prime passerelle con i giubbotti della Protezione civile, con gli stivali nel fango e con l'elicottero, ma adesso sembra che il tema sia stato accantonato e non se ne ricordi tantissimo. Ci penserò continuamente interventi per ricordare quello che succede in Emilia-Romagna. Siete riusciti finalmente, dopo sessanta giorni, a nominare un commissario della ricostruzione e direi: meglio troppo tardi che mai. L'evento del 3 maggio, poi ripetutosi il 16 e 17 maggio e arrivato fino al 29, ha dato un'errata percezione di quello che sta succedendo. Le ruspe che stanno lavorando sull'emergenza sono le stesse che devono lavorare in sinergia con il il tema della ricostruzione. Un commissario alla ricostruzione che arriva dopo sessanta giorni ha quasi impedito di portare avanti i lavori in questo momento. Ho girato l'entroterra in questo periodo, ci sono tantissimi Comuni che sono in forte difficoltà. Abbiamo avuto più di mille frane e penso che quest'Assemblea non si renda conto di quello che è successo: alcune di esse sono talmente gravi che non saranno neanche più ripristinate e ci sono Comuni isolati.

completamente vuoti. Come ha detto la nostra Presidente del Consiglio, avete raschiato il fondo del barile per dare uno stanziamento economico ed è una cosa inaccettabile, perché proprio

Il sistema sanitario non è stato in grado di garantire su tutto il territorio nazionale un'assistenza uniforme per quantità e qualità. Questo monito del 2022 non proviene da una forza di opposizione in cerca di uno scontro politico con la maggioranza, bensì dalla Corte dei conti. La riforma del Titolo V ha inaugurato una stagione nuova per molte materie statali, tra cui la sanità, parcellizzate in tante «repubbliche cisalpine». L'Italia necessita di un'unica cabina di regia: lo Stato, tanto caro a Montesquieu, eliminato dalla bicamerale di D'Alema e Berlusconi. La sperimentazione del modello di gestione regionale della sanità è fallita, infatti si è avuto un incremento della spesa improduttiva, cioè quella non legata alla salute dei cittadini. Presidente, onorevoli colleghi, come medico, prima che come cittadina, sostengo che l'approccio alla medicina dev'essere olistico; bisogna cioè valorizzare, oltre alla diagnosi e alla cura, la prevenzione e la qualità della vita. L'esperienza della pandemia ha acceso un riflettore sulle molteplici criticità che si annidano nella frammentazione gestionale della sanità, che ha generato territori di serie A e territori di serie B, non solo tra Nord e Sud, ma nelle stesse Regioni del Settentrione come ad esempio, in Lombardia, Bergamo e Brescia. Durante la pandemia i medici si sono trovati a dover scegliere se intubare un anziano o un ragazzo, perché in quei territori non vi erano più posti letto. Questo è avvenuto perché dal 2001 sono stati fatti continui tagli alla sanità, inoltre si è proceduto ad assegnare, non solo meno risorse, ma, utilizzando l'artificio della spesa storica, si è creata una sperequazione tra le Regioni settentrionali e quelle meridionali e così nel 2018 la Liguria ha incassato quasi 2.600 euro per cittadino, mentre la Calabria solo 2.200. Presidente, onorevoli colleghi, ovviamente non intendo puntare il dito contro le Regioni che hanno ottenuto più fondi, ma mettere in evidenza che il sostegno statale dev'essere equo, cioè *pro capite* per tutte le Regioni, e se c'è un capitolo di spesa che non bisogna mai tagliare è quello Consideriamo altresì che ben sette Regioni, tutte del Centro-Sud, sono finite soggette alla disciplina dei piani di rientro, per cui i commissari hanno dovuto limitare l'accesso alle cure a milioni di cittadini, così assistiamo a lunghe liste d'attesa e al triste fenomeno della mobilità sanitaria. Pertanto, chi non può permettersi il viaggio della speranza è destinato a soccombere. Noi del MoVimento 5 Stelle lotteremo contro questo provvedimento, continuando a difendere una sanità equa, gratuita e accessibile a tutti. La sanità è patrimonio universale e non appannaggio di pochi privilegiati. Se necessario, utilizzeremo anche la strada referendaria. Signora Presidente, prendo la parola per affrontare un tema importante che riguarda migliaia di italiani all'estero. L'Italia in passato ha fatto ricorso allo strumento delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale per dare un quadro di certezza normativa alle questioni di natura previdenziale e assistenziale. La finalità degli accordi di sicurezza sociale è quella di garantire la parità di trattamento di lavoratori e pensionati che si spostano dall'uno all'altro Paese contraente, oltre che la totalizzazione dei periodi contributivi. L'Italia, come sappiamo, storicamente Paese di emigrazione, necessita forse più di qualsiasi altro nel mondo dell'efficacia di tali accordi bilaterali di sicurezza sociale, che consentono quindi ai lavoratori italiani emigrati e ai lavoratori stranieri immigrati in Italia di attivare il meccanismo della totalizzazione dei contributi versati nei Paesi contraenti. Eppure il sistema di tutela previdenziale in regime internazionale non è completo, poiché numerosi Paesi di emigrazione italiana sono rimasti esclusi. Fra questi vi è il Messico, con il quale l'Italia ha sviluppato nel tempo importanti relazioni e dove risiedono oltre 25.000 cittadini italiani iscritti all'Anagrafe italiani residenti Con il Messico l'accordo è in vigore dal 1977, ma è applicato soltanto ai cittadini italiani rimpatriati, titolari quindi di pensione messicana, mentre per gli italiani residenti in Messico che hanno maturato contributi pensionistici in Italia l'erogazione di un'eventuale pensione praticamente non avviene. È evidente come tali accordi siano anacronistici e anche limitatori nei confronti dei rapporti solidissimi Il nostro Paese, il tredicesimo fornitore del Messico, è il secondo *partner* commerciale europeo dopo la Germania. I benefici che deriverebbero dalla vigenza di tali accordi internazionali sarebbero fruiti non solo dai lavoratori interessati, ma anche dalle imprese italiane, che sarebbero in grado in grado così di aumentare la propria competitività sul piano internazionale. Era il lontano 2016, signora Presidente, quando presentai alla Camera un atto di sindacato ispettivo per chiedere quali iniziative urgenti si intendessero adottare per completare il quadro di tutela previdenziale in regime internazionale con la stipula di una convenzione di sicurezza sociale con il Messico, dove vive una vasta e importante comunità di cittadini italiani. Le risposte di allora furono insoddisfacenti. Nel frattempo, ho indirizzato altre interrogazioni ai vari Ministri, ma le risposte sono sempre state altrettanto insoddisfacenti. Mi chiedo, e concludo, signora Presidente, quale sia la politica del Governo in relazione alla tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori italiani in Messico e dei lavoratori di tale Paese Paese in Italia titolari di regolare permesso o carta di soggiorno. Bisogna intraprendere immediatamente delle iniziative per completare il quadro di tutela previdenziale internazionale, stipulando una convenzione di sicurezza con il Messico. Sono troppi gli interessi e troppo poche le risposte positive che stiamo dando ai cittadini italiani nel mondo.